desidero comunicare all'Assemblea che alcuni Gruppi politici hanno già esaurito il tempo a loro disposizione e che altri sono sulla soglia dell'esaurimento. ricordo che a conclusione della Conferenza dei Capigruppo è stato introdotto il contingentamento dei tempi con l'obiettivo - reso anche esplicito - di pervenire, nella giornata odierna, alla conclusione dei nostri lavori e al voto

Per i Gruppi che hanno esaurito i tempi di discussione naturalmente il diritto ad intervenire per illustrazione o dichiarazione di voto non c'è.

l'illustrazione di eventuali residui emendamenti e per esercitare il diritto della dichiarazione di voto finale. Ieri la seduta ha avuto un andamento imprevisto in quanto ci si è soffermati su un argomento delicatissimo quale quello relativo alla realizzazione o meno del ponte sullo Stretto e, in particolar modo, sulla presentazione di un ordine del giorno, a firma dei Capigruppo della Casa delle Libertà, che impegnava il Governo a non ritenere il decreto-legge che trasferisce i fondi dalla società Stretto della possibilità che l'opera sia realizzata con altri fondi; quindi, un impegno politico di un'assenza di pregiudizialità contraria alla realizzazione di quest'opera, anche se con fondi privati, con fondi europei, ma non con fondi statali, quale era la volontà del Governo. Questo è un ordine del giorno importantissimo sul quale ci siamo soffermati. Abbiamo preso atto di una volontà pregiudizialmente avversa da parte del Governo e della maggioranza alla realizzazione di quest'opera senza se e senza ma. Questo ci ha impegnato per alcune ore. Detto questo, Presidente, sulla sua osservazione relativa al tema del richiamo al Regolamento, vorrei ricordare che

si chiede di aggiungere «privilegiando la realizzazione di infrastrutture trasportistiche di accesso e connessione al ponte ». Anche in questo caso è nota la posizione di chi come noi da tempo è contrario al ponte. Ne ha fatto oggetto di una battaglia politica anche con le forze ambientaliste in Calabria e in Sicilia e tuttavia, ecco la questione politica, beneficio dell'Aula che nelle Commissioni riunite quinta e sesta i due relatori hanno predisposto un ordine del giorno che sintetizzava analoghi ordini del giorno da noi presentati che ovviamente prevedevano, secondo quanto indicato dal decreto, la destinazione delle risorse finanziarie nella misura del 90 per cento per le infrastrutture in Calabria e in Sicilia per cento per interventi di tutela dell'ambiente e della difesa del suolo nell'ambito della ripartizione già prevista 70 e 30 per cento. Allora, non ci prendiamo in giro: qui il tema non è solo metodologico. Certo che abbiamo privilegiato il confronto in Commissione sugli ordini del giorno accogliendone anche alcuni dell'opposizione, ma il problema è un altro. Quando nell'emendamento si parla di privilegiare la realizzazione delle infrastrutture di accesso al ponte, si dà per scontato che la scelta fatta, che comunque vede il ponte assolutamente non prioritario e comunque conseguente ad altri interventi, è una scelta che non si condivide. Ecco perché il nostro non è un artificio formale, non è una questione solo tattica legata alla scelta di non modificare il decreto; su questo punto c'è un dissenso strategico, il dissenso sul fatto che privilegiamo le infrastrutture trasportistiche di sviluppo, sia in Calabria che in Sicilia. Ecco perché siamo contrari all'emendamento in

Presidente, avendo ascoltato il collega del Gruppo di Rifondazione Comunista mi sembra che sia lapalissiano nel suo ragionamento un argomento che però la coalizione che sostiene il Governo in qualche modo nega, perché dovrebbe contraddire se stessa e i programmi precedenti. Fondamentalmente, nella sua valutazione c'è l'esclusione assoluta del ponte, mentre voi avete detto come Governo che l'opera è semplicemente non prioritaria e potrebbe realizzarsi con tempistiche e modalità diverse. La scelta di questo emendamento tentava di tenere insieme ambedue le questioni, perché le opere di connessione trasportistica sono comunque fungibili, è stato spiegato ampiamente dai tecnici: sono fungibili con un sistema che non preveda il ponte, ma sono utilizzabili anche senza ponte. Ma la scelta ideologica è talmente forte da escludere anche il buonsenso.

Signor Presidente, ho chiesto la parola su questo emendamento che ho fatto mio non essendocene altri su cui poter intervenire - per parlare della normativa riguardante un ulteriore aggiustamento alla materia dell'editoria, materia molto delicata, sulla quale

decreto-legge n. 223 del luglio scorso. La questione riguarda in particolar modo l'editoria dei partiti politici. Nel decreto n. 223, precisamente all'articolo 20, si è proceduto ad un ritocco che interessava particolarmente quella editoria di partito che aveva subito, nel corso dell'ultima consultazione elettorale, qualche punto di incidenza. Mi riferisco soprattutto a quei Gruppi parlamentari, come quello dell'Ulivo, per esempio, che si era costituito attraverso l'unione di due partiti (la Margherita e i DS), i quali avevano organi di partito che percepivano

aggiustato il metodo seguito per l'elargizione di questi contributi sulla base della nuova situazione che si è venuta a creare con le elezioni del 9 aprile. non si è tenuto conto, e non si tiene conto nemmeno in questo provvedimento legislativo, che ci sono nuove realtà politiche, nuovi Gruppi costituitisi che non hanno potuto ereditare i requisiti soggettivi, precedentemente stabiliti con la normativa vigente applicabile, e che non potrebbero usufruire dei benefici previsti dalla normativa sull'editoria a favore degli organi di partito. Ebbene, così come è stata aggiustata la normativa

ritengo che, attraverso il ritiro di questo emendamento e la presentazione di un ordine del giorno, che mi accingo a presentare (sto finendo di redigerlo), si possa dare un indirizzo al Governo in modo che, con il regolamento che si accinge

nuova situazione che si è venuta a creare dopo il 9 aprile con il sistema proporzionale, con nuovi Gruppi e nuove realtà, ridefinendo ridefinendo anche i requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici. Di questo è importante tener conto. Oggi infatti vi sono organi di partito - tutti possiamo verificare

presenti 318, votanti 317, maggioranza 159, favorevoli 162, contrari 164, astenuti 1. **Il Senato approva.**

Dichiaro aperta la votazione. presenti 318, votanti 317, maggioranza 159, favorevoli 162, contrari 164, astenuti 1. **Il Senato approva.**

I commi 124, 125 e 127 nascono dal caos determinato dalla mancanza di approvazione del disegno di legge Bonaiuti e dall'altalenante modalità di determinazione dei contributi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con le modifiche indicate si evitano sperequazioni a favore di alcune imprese a danno di altre, prevedendo la media dei costi abrogata dal 2002 senza soluzione di continuità, mentre la formulazione originaria prevedeva che tale sistema fosse adottato solo per gli esercizi 2002-2003 e 2006. Pertanto, per equità, chiediamo l'approvazione di questo emendamento.

presenti 318, votanti 317, maggioranza 159, favorevoli 162, contrari 164, astenuti 1. **Il Senato approva.**

Con l'emendamento in oggetto si destina il contributo unicamente ai giornali editi all'estero in lingua italiana, piuttosto che ai giornali editi all'estero in lingua straniera. Quindi se vogliamo promuovere la informazione italiana è giusto che sia fatta in lingua italiana.

prevede una riserva di legge per quanto riguarda qualsiasi intervento che regolamenti e disciplini gli enti di ricerca. Voglio qui rapidamente anche ricordare l'appello del Consiglio universitario nazionale, che ha chiesto ai parlamentari di scongiurare i gravi rischi che deriverebbero alla ricerca scientifica

CGIL, CISL e UIL addirittura chiedono di cassare queste norme, perché paventano un irreversibile degrado di un patrimonio di risorse umane scientifiche insostituibili. L'Associazione nazionale professionale per la ricerca della funzione pubblica dice lo stesso; anzi, con toni molto determinati, chiede che venga rispettata la Costituzione e che venga evitato questo progetto di riordino, che ha per unico scopo quello di creare nuovi strapuntini e nuove poltrone, infischiandosene dell'autonomia della ricerca universitaria.

una prima votazione per l'abrogazione dei commi 159, 160 e 161 ed una seconda votazione per l'abrogazione del comma 162.

di questo ramo del Parlamento in ragione di incarichi istituzionali precedenti o per merito e ai membri della Commissione affari costituzionali.

persona. I commi precedenti, infatti, prevedono che i dirigenti di istituzioni statali provenienti dal privato abbiano diritto ad essere risarciti per la durata dei contratti in essere, se revocati; i dipendenti pubblici non hanno nemmeno diritto al risarcimento. Il comma 162 riguarda un solo dirigente che proviene dal privato e che verrebbe mandato a casa, ove venisse presa questa posizione, senza nemmeno il risarcimento. È evidente che qualunque ricorso darebbe

nulla da eccepire, anche se magari potremmo domandarci se uno *spoils system* così vasto, in qualche modo, non possa inficiare le strutture ministeriali, e in qualche modo vanificare la legge Bassanini che, ricordo,

non stava assolutamente in piedi, perché andava ad interrompere contratti che avevano, evidentemente, un'assoluta validità dal punto di vista civilistico; inoltre, affermava che i contratti erano nulli, una bestialità giuridica enorme. La Camera ha cercato di

del contratto. Ciò significa che vi saranno dirigenti che percepiscono somme anche notevoli, superiori ai 100 milioni all'anno

Sul gazzettino di Prodi, meglio noto come «Corriere della Sera», abbiamo visto sproloquiare addirittura sulla possibilità che questo Governo potesse licenziare i lavoratori nullafacenti,

Ricordo - ministro Mastella, mi rivolgo a lei perché è presente - che questa è una norma che dà una possibilità e non impone certo l'obbligo di fare ciò. Posso testimoniarle, perché li conosco uno per uno, che i dirigenti del suo Ministero sono persone assolutamente valide dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista etico, nel senso che interpretano perfettamente la legge Bassanini che dà al Ministro la possibilità,

Lei sa che cosa ho fatto, al di là del dovuto? Io sono tra i pochi - credo - che ha realizzato una congiunzione tra chi c'era e chi oggi presiede questo Dicastero. Se vuole la mia opinione,

presenti 318, votanti 317, maggioranza 159, favorevoli 162, contrari 164, astenuti 1. **Il Senato approva.**

Noi proponiamo che siano confermate ove non revocate: questo vuol dire che, almeno, vi sia una motivazione se si manda via una persona, persona, lo sforzo di fornire una motivazione al fatto che si manda via una persona debba essere compiuto anche da un Governo che ha scoperto l'America da quando...

questa roba provoca una valanga di ricorsi. Credo che il giorno dopo la sentenza della Consulta, l'acronimo di Tommaso Padoa-Schioppa, TPS, diventerà «Tanto Passa Subito», perché così non si può andare avanti!

Presidente, le chiedo licenza di venti secondi in più. Colleghi, prima ho tentato di esporre le ragioni dell'ingiustizia determinata dal comma 162, che è una norma contro una persona. Stiamo cercando di rimediare nella filosofia proposta dalla maggioranza, che prevede che i dirigenti delle agenzie possano essere mandati a casa; con questo emendamento s'include almeno l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, per la quale era stato previsto un comma a parte, con lo stesso trattamento riservato dal comma precedente alle altre agenzie. È un atto di giustizia per evitare una legge contro una persona, colleghi! Credo che anche coloro i quali in Commissione affari costituzionali hanno espresso parole per evitare disparità di trattamento si debbano mettere la mano sulla coscienza per evitare un'ingiustizia di una legge contro una persona sola.

Presidente, molto brevemente, abbiamo presentato questi emendamenti per dare anche la possibilità al Governo di ripensare e rivedere questa posizione assunta nel decreto-legge fiscale nel quadro generale della manovra finanziaria. Ci rendiamo conto che ci sono delle esigenze del Governo di approvare immediatamente questa legge; quindi, facendo politica, comprendiamo comprendiamo le ragioni degli altri. Però, c'è la legge finanziaria. Chiediamo ai rappresentanti del Governo, ai relatori, di poter in qualche modo orientare la legge finanziaria in maniera che si venga a lenire parte di questo di questo aspetto mortificante per la pubblica amministrazione contenuto in questa norma. Chiediamo ciò al Governo: avete ancora a disposizione la legge finanziaria, in quella sede potete fare le correzioni che abbiamo indicato in maniera chiara e precisa.

Presidente, siamo ancora sul tema riguardante l'Agenzia per i servizi sanitari. L'Assemblea ha deciso che si può mandare via una persona senza risarcimento, anche se viene dal privato: così è stato deciso e io mi inchino alla volontà dell'Assemblea.

auspicando, anche in maniera molto forte (e io sono d'accordo con loro), il rigore della finanza pubblica e che oggi credono di salvarsi l'anima non votando contro questi emendamenti, che in qualche modo sono a favore del rigore della finanza pubblica, ma semplicemente astenendosi. Ebbene, sappiamo tutti che il voto di astensione in Senato

Rispetto ad una situazione di favore, che prevedeva i sindacati in una condizione privilegiata, ho previsto di estendere questa normativa anche agli enti benefici, alle ONLUS, soggetti sociali, istituzioni autorizzate e associazioni culturali. Mi sembra una richiesta di buonsenso, anche se ritengo che tale apertura sia poca cosa rispetto alla complessità di questo provvedimento di accompagnamento.

Presidente, credo che l'Aula debba riflettere per un momento su questo ordine del giorno, che presenta molte ambiguità

di un passaggio generazionale delle imprese anche nell'ambito familiare, prevede una franchigia per i trasferimenti a favore dei fratelli ovvero di persone

«a prevedere l'applicazione della franchigia ai trasferimenti a favore di altri soggetti diversi dai parenti in linea retta, a partire dai fratelli.». Credo che questa formula ambigua richieda anche un parere da parte del Ministro della giustizia, oggi presente in Aula, rispetto alle tante parole spese in favore della famiglia

a prevedere l’applicazione della franchigia ai trasferimenti a favore di altri soggetti diversi dai parenti in linea retta, a partire dai parenti in linea collaterale di secondo grado; a

cui si dice: «a prevedere l'applicazione della franchigia ai trasferimenti a favore di altri soggetti diversi dai parenti in linea retta».

ho colto la preoccupazione del collega Eufemi. Questa formula potrebbe indurre a ritenere che ci sia un invito al Governo ad estendere le norme di franchigia anche a soggetti che non siano affatto parenti.

parenti diversi da quelli previsti, che siano comunque parenti, ovvero che facciano parte della famiglia legittima e non di altre situazioni che potrebbero essere ricomprese.

venga estesa ed ampliata. È una richiesta di generalizzazione della franchigia.

presenti 318, votanti 317, maggioranza 159, favorevoli 162, contrari 164, astenuti 1. **Il Senato approva.**

un capoluogo d'Italia, di questo sciagurato Paese, che non è ancora collegato con la rete autostradale nazionale. C'è una Provincia che è la prima Provincia italiana per la prima Provincia italiana per il lavoro, quindi con il più basso tasso di disoccupazione e la più alta percentuale di partite IVA (per ogni tre abitanti c'è una partita IVA), che però non ha una strada: non dico dieci strade, ma una sola strada di grande comunicazione.

dei nuovi criteri voluti sciaguratamente dal ministro Di Pietro, quindi, impedirà di fatto la realizzazione di quest'opera. L'unico modo per poter dare speranza a quella Provincia, a quei cittadini, a quelle popolazioni

Le ragioni sono state ampiamente illustrate; ieri il senatore Martinat è intervenuto sull'impedimento essenziale per la realizzazione di quest'opera. Con questo intervento, credo di poter chiedere anche

complesso, a cui hanno partecipato tutte le forze politiche, i partiti, le categorie economiche e tutti gli enti per

come sanno tutti i componenti della Commissione infrastrutture, che la vicenda dei tratti autostradali Asti-Cuneo e Brescia-Bergamo-Milano è scandalosa perché il Governo con ciò rinuncia all'apporto di importanti capitali privati in un Paese in cui le risorse pubbliche sono sempre più carenti.

poiché essa si riferisce alla limitazione dell'attuazione della normativa di cui ci stiamo occupando alla fattispecie indicata nella premessa. Un ordine del giorno non può ovviamente impegnare il Governo a limitare l'attuazione di una norma di legge. Pertanto, eliminando la parte che ho indicato, si può pervenire ad un parere favorevole, perché in tal modo si rileva che il problema posto dai presentatori

dal Governo. Peraltro, in Commissione su questo punto abbiamo fatto un lavoro molto approfondito pervenendo alla formulazione di un ordine del giorno, approvato in Commissione, che impegna il Governo a una riflessione su questa materia. Quindi, l'ordine del giorno in tal modo riformulato sosterrebbe anche l'indicazione contenuta nell'ordine del giorno di cui ho detto.

senatore Barbato,

È un punto che per i relatori e, suppongo, per il Governo non è accettabile perché non si può approvare, come stiamo facendo, una norma di legge e poi impegnare il Governo a non applicarlo ad un istituto, seppur prestigioso, come il

affidata allo strumento legislativo e non regolamentare, come previsto dai commi 143, 144 e 145 noi relatori abbiamo presentato insieme ad altri colleghi, afferma tale principio, quindi recepisce, seppure con una formulazione più sintetica, la sostanza dell'ordine del giorno

riproducendo esattamente il parere espresso dalla 7a Commissione, approvato all'unanimità. Non vi dovrebbe quindi essere alcun problema da parte dei presentatori ad aderire alla formulazione dell'ordine del giorno G2.800, così come

Vorrei sottolineare che abbiamo lavorato con assoluta funzionalità.

la invito a riflettere mi sembra chiara. Qui non stiamo modificando una deliberazione già formalizzata e approvata dall'Aula,

Presidente, come si può scrivere in un ordine del giorno che si impegna il Governo a fare una disposizione contraria alla legge di contabilità?

Pur tuttavia, un esame attento dell'ordine del giorno G2.800 porta a concludere che nel testo non si afferma quanto testè detto dal senatore Ferrara, perché si legge: legge: «impegna il Governo a procedere quanto prima al riordino degli enti di ricerca menzionati a mezzo di legge delega e conseguenti decreti legislativi al fine di promuovere l'autonomia statutaria degli enti medesimi». Questa formulazione, signor Presidente, è esattamente riproduttiva

Dopodiché si dice: «ad affrontare il problema già con la prossima legge finanziaria», non si dice di inserire nella legge finanziaria una legge delega; il che è problema diverso. Quindi, mi sembra chiaro che l'obiezione del senatore Ferrara, a parere del relatore, può ritenersi ampiamente superata.

sicuramente, la maggioranza hanno compreso il pasticcio in cui sono incorsi nell'accettare i commi 143, 144 e 145. la maggioranza si è fatta scippare completamente dall'onorevole Mussi, ministro dell'università, la riforma degli enti di ricerca. Sono qui presenti personaggi che hanno fatto la storia del Paese, i quali sanno benissimo che i ricercatori vogliono certezze. Ebbene, con questo decreto le certezze non ci sono.

Allora dovete chiedere: caro Mussi, ci fai la gentilezza di non applicare questa legge? Solo questo è il modo per comprendere l'ordine del giorno. Pertanto, sono contrario all'ordine del giorno non tanto per l'ordine del giorno in sé, ma per l'errore

intervengo brevemente per rispondere al relatore, che mi ha rivolto un invito. Innanzitutto, apprezzo lo spirito di questo ordine del giorno e il fatto che sia un passo in più. Vorrei però brevemente ricostruire la vicenda, perché su questo ordine del giorno c'è stato un invito, venuto da illustri esponenti della maggioranza, a ritirarlo e a riformularlo. Credo che la riformulazione, tra l'altro, abbia aggiunto ricchezza a quest'ordine del giorno, introducendo in particolare un elemento:

al Governo affinché non lo applichi per l'ente più prestigioso ed importante, per cui la lesione dell'autonomia sarebbe, in qualche modo, un *vulnus* aggravato

Il Governo non ha messo la fiducia su questo decreto-legge: onore al Governo. La maggioranza in quest'Aula ha rifiutato il confronto con l'opposizione. Non ha accettato nessun emendamento dell'opposizione, in alcuni casi sapendo di fare una cosa sbagliata, persino vergognosa: ci ha detto che per disciplina di partito votava cose che sapeva essere sbagliate. Attraverso gli ordini del giorno si tenta in qualche modo di recuperare e di mettere a posto la propria coscienza. Anche questo non si può fare compiutamente perché non c'è sufficiente coraggio. Il dialogo, che sarebbe stato possibile nella discussione di questo disegno di legge, è stato rifiutato Più di una volta vi abbiamo sentito dire: è vero, avete ragione, nella finanziaria cambieremo. Ma se una cosa è giusta, perché non farla qui e ora?

Detto questo, ritengo che tale ordine del giorno sia insoddisfacente per due aspetti: in primo luogo, perché introduce un giudizio politico, cioè chiede che quanto prima venga effettuato il riordino degli enti di ricerca. Noi non siamo d'accordo che venga effettuato quanto prima, perché su tale riordino politicamente non concordiamo. Quindi, innanzitutto, chiederei di eliminare le parole «quanto prima». Inoltre, si chiede che questo

colpo di mano, dato che nella finanziaria non c'è la possibilità di sviluppare un adeguato dibattito fra le forze politiche. Per votare questo ordine del giorno, chiedo che lo si riformuli come segue: «impegni il Governo ad abrogare i commi 143, 144 e 145, prevedendo che il riordino degli enti di ricerca avvenga a mezzo di apposita legge delega». Ritengo che una formulazione di questo tipo, che non fa riferimento alla finanziaria, in cui non c'è il riferimento all'urgenza di una riforma, potrebbe essere tranquillamente accettata.

2). Vorrei inoltre segnalare che il problema della costituzionalità ha formato oggetto delle pregiudiziali e quindi è una materia che credo sia stata metabolizzata dall'Aula.

questa materia è oggetto di riserva di legge a norma dell'articolo 33 della Costituzione, ma la stessa formulazione del ricorso a regolamenti di delegificazione - così come fatta in questi commi e come rilevato con grande serietà dal Servizio studi del Senato - è assolutamente impropria, dal momento che mancano molti degli elementi affinché il Governo possa far riferimento all'articolo 17 della legge fondamentale in materia.

Presidente, il problema posto dai due ordini del giorno in esame è un problema vero e reale: è la ragione per la quale avevo sottoscritto

anche aggiungere una considerazione a quanto veniva testé detto dal collega Buttiglione. Vede, Signor Presidente, abbiamo visto di tutto durante l'approvazione di questo decreto-legge. Ci sono state anche Commissioni, per esempio la Commissione agricoltura cui appartengo,

sono poi comportati in Aula in maniera assolutamente opposta rispetto alla condizione da loro stessi votata. Abbiamo visto veramente di tutto: vi è stata una blindatura assoluta e una totale sordità da parte della maggioranza nei confronti delle ragioni dell'opposizione.

leggi delega e decreti legislativi a meglio definire e garantire l'autonomia statutaria degli enti culturali vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.

Dichiaro aperta la votazione.

Non capisco le ragioni per le quali il relatore e il Governo abbiano espresso parere contrario. Abbiamo semplicemente rappresentato la gravissima crisi delle Ferrovie dello Stato. Abbiamo chiesto che venga reso pubblico il bilancio consolidato delle Ferrovie, che ad oggi ancora non è disponibile, e l'ingegner Moretti è venuto nei giorni scorsi a chiedere ingentissime risorse al Parlamento. Mi domando se questo è un atto di lesa maestà. Chiediamo di rivedere la struttura societaria riducendo le società controllate, chiediamo di eliminare ogni area di spreco, compreso il finanziamento del veltronismo che è avvenuto da Trenitalia, una società in perdita e che quindi viene pagata dalla fiscalità generale. Queste sono le ragioni che mi inducono a chiedere la votazione dell'ordine chiedo un minuto di tempo; credo di averne diritto perché parlo in dissenso dal mio Gruppo, immaginando che esso voti l'ordine del giorno G2.115. Non voterò questo ordine del giorno e intendo chiarire i termini della questione, perché non condivido l'affermazione che le Ferrovie siano in una grave situazione finanziaria. Questa storia della Ferrovie in stato di pre-fallimento è stata creata dall'ingegner Moretti che andando alla trasmissione «Ballarò» ha fatto questa affermazione, ripresa poi dal «Corriere della Sera». Peccato che l'ingegner Moretti nei mesi scorsi ha trasmesso al ministro Padoa-Schioppa una documentazione dalla quale emerge che nei cinque anni del Governo Berlusconi le Ferrovie hanno avuto ben 27 milioni di euro per investimenti e risorse nel capitale di esercizio. Durante i Governi Prodi, D'Alema e Amato le Ferrovie hanno avuto meno di 9 milioni di euro. Questa storia quindi non

perché da anni le Ferrovie dello Stato non hanno chiarito un punto fondamentale. Nel 1999 fu consentito alle Ferrovie dello Stato di usare finanziamenti pubblici in conto capitale nel conto corrente e, così, per magia, apparve un risanamento finanziario del conto economico dello Ferrovie dello Stato. In quel momento, cioè sette anni fa, le Ferrovie, spostando investimenti dal conto capitale al conto economico, risanò apparentemente e aritmeticamente i conti delle stesse Ferrovie, con l'impegno di rimettere in finanziamento per investimenti attraverso le risorse auto finanziate delle Ferrovie. Quindi, prima di decidere qualunque ulteriore finanziamento pubblico alle Ferrovie, l'azienda ha il dovere di chiarire al Parlamento e al Governo che fine hanno fatto quei fondi e come intende recuperarli e riportarli nella contabilità degli investimenti.

presenti 318, votanti 317, maggioranza 159, favorevoli 162, contrari 164, astenuti 1. **Il Senato approva.**

parte che recita: «che la rappresentanza parlamentare conseguita alle elezioni politiche, con la costituzione di Gruppi parlamentari sia alla Camera che al Senato, devono essere ritenuti

«impegna il Governo: a rivedere la disciplina della materia dei contributi per l'editoria degli organi di partito (giornali quotidiani, periodici, giornali telematici, agenzie, radio e TV); ad integrare, eventualmente, la vigente normativa nel senso di cui al presente ordine del giorno». Si è resa necessaria tale rivisitazione di tutto l'ordine del giorno al dine di ottenere il più ampio coinvolgimento delle forze politiche

ne ha letto uno diverso da quello distribuito, vorrei essere certo che sia scomparso, nell'ultima stesura, qualunque riferimento alla rappresentanza parlamentare e spiego brevemente perché.

polemica. Questa non è una legge. Non possiamo dare l'impressione che crediamo che la rappresentanza politica sia esclusivamente quella parlamentare.

ogni riferimento alla rappresentanza parlamentare riferita ai Gruppi parlamentari. Siccome potrebbero mutare, è necessario evitare che una legge ingabbi l'evoluzione del quadro politico.

presenti 318, votanti 317, maggioranza 159, favorevoli 162, contrari 164, astenuti 1. **Il Senato approva.** *(Generali

molto rapidamente, anche se queste sono le condizioni meno opportune per esprimere qualche considerazione.

della maggioranza, ma quale rappresentante del Senato della Repubblica, perché credo che abbiamo finalmente innovato il nostro modo di procedere nei lavori del Senato. Senato. Il non aver posto la questione di fiducia ha infatti dato la possibilità al Senato di essere davvero la Camera alta: i senatori si sono sentiti nell'esercizio delle loro funzioni e nella pienezza dei loro poteri. Penso che abbiamo scritto una pagina significativamente bella dei lavori del Senato in questa legislatura. Auspico e mi auguro che con la presidenza del presidente Marini altre pagine di questo tenore si possano scrivere, nel senso che il primato della politica e del Parlamento vengano sempre più esaltati nella conduzione

Lasciando ad altre sedi l'esame, che peraltro è già stato approfonditamente dibattuto e risolto, sui doveri e sui diritti dei senatori a vita, a me preme soltanto fare presente una cosa, rivolgendomi senatori che hanno fatto riferimento alla non esistenza del mandato popolare dei senatori a vita e quindi ad un loro incidere nelle scelte democratiche del Paese non essendo forniti, alla base, del titolo che consente a tanti altri senatori, alla stragrande maggioranza del Senato, di incidere. A me preme soltanto ricordare che buona parte di questi senatori a vita, che oggi siedono, in virtù di una norma costituzionale - e *de iure condito* non potrebbe essere altrimenti - è approdata negli anni scorsi, sugli scranni parlamentari, sulla base di suffragi che hanno visto decine e decine di migliaia di voti che li hanno portati ad essere deputati o senatori. Pensare che questi nostri colleghi non siano muniti del titolo per rappresentare gli italiani è offensivo unicamente ed esclusivamente per coloro che pensano ciò. Non credo di dovere aggiungere altro.

mi associo a quanto è già stato detto dal collega Formisano riguardo ai senatori a vita.

né è possibile indugiare oltre. Infatti, lo sappiamo, questo collegato non è oltremodo differibile, in primo luogo, per ridefinire la finanza pubblica; in secondo luogo, perché le disposizioni contenute saranno valutabili a lungo termine; infine, come ho sostenuto dall'inizio, perché ci incombe l'obbligo di iniziare l'esame della legge finanziaria vera e propria, preludio di altre tappe importantissime del nostro percorso di legislazione. Giocoforza é basilare è provvedere celermente all'approvazione; mi sento in dovere di rilevare che, nel merito della questione, il Governo ha cercato di confrontarsi produttivamente con tutte le parti politiche e con le categorie interessate nello specifico della manovra fiscale. Laddove si è potuto influire, si è influito poco. Siamo certi che questo ramo del Parlamento si farà promotore di interventi incisivi nei lavori di esamina della legge finanziaria. Bisogna aggiungere, altresì, che i contenuti del decreto hanno imposto, per necessità di celere conversione, di procedere in tempi di esame molto ristretti, tant'è che anche i miei lavori hanno subito freni a fronte dell'interesse superiore che è in gioco. Interesse che va verso obiettivi di contenimento definitivo dell'economia sommersa, verso la definizione di nuove entrate e tagli di spesa, verso, cioè, misure specifiche per ripartire equamente il carico fiscale e consentire all'Italia di stare ai tempi. Certamente non ho rinunciato a lottare per gli interessi di cui sono portavoce e ho sopperito all'esclusione degli emendamenti proposti, compulsando il Governo ad impegnarsi in tema di successioni e donazioni, per evitare aggravi di costi e adempimenti a carico di soggetti con disabilità ed in tema di sicurezza dei territori per tentare di evitare la soppressione del RID. In ogni caso, sono consapevole del valore di questo decreto che va oltre il tentativo di rimozione dell'evasione fiscale e compie l'ulteriore sforzo di mitigare le misure limitative a carico del ceto medio, al fine di non vessare pesantemente imprenditori e professionisti. Ciò vuol dire che il Governo ha dimostrato di avere a cuore la stragrande maggioranza degli italiani, che sono onesti e producono, quella parte di società che è produttiva e che ha bisogno di essere tutelata. Nel concludere, perciò, ribadisco che il provvedimento è di fondamentale importanza, a garanzia dell'economia e del rilancio del nostro Paese. Per questo abbiamo scelto con convinzione di votare positivamente per la conversione in legge del decreto-legge n. 262. *(Applausi

Naturalmente, gli interventi precedenti hanno richiamato alcune pagine del dibattito che ha circondato il decreto fiscale, fornito ai senatori in edizione panino con la finanziaria, nel senso che l'uno precede l'altra e trasmette al Paese i primi gemiti del lamento prolungato che accompagnerà il varo di queste misure. misure. Il decreto fiscale rievoca, infatti, fantasmi che, pur con i limiti che tutte le azioni di Governo hanno, il quinquennio precedente aveva in qualche modo allontanato. Torna la tassa di successione, che, si dice, riguarda solo i patrimoni che superano un milione di euro. Ma chi oggi guarda gli annunci immobiliari,

Inserti di quotidiani importanti definiscono il nostro tempo «il secolo dei centenari». Il centenario che ci lascia e se ne va magari ha un appartamento in centro che ai suoi tempi era una casa popolare, mentre adesso vale due milioni di euro. Probabilmente, lasciandolo agli eredi, non è lieto di carburare e rifornire il Governo Prodi di un 6 per cento, estensibile all'8 per cento, se ci sono circostanze che fanno ritenere quest'unico bene una ricchezza. Vorrei altresì ricordare le dichiarazioni del ministro Padoa-Schioppa - diffido sempre di chi ha troppi cognomi, perché l'aura di nobiltà dà licenza di libertà assoluta nell'eloquio - poiché, a margine di un convegno,

Ovviamente, chi si appresta a tirare l'ultimo bottone della cinghia - se può farlo - per alimentare una manovra finanziaria ben diversa, si domanda perché sia richiesto il giro di vite fiscale che questo decreto annuncia come il ritmo di un tamburo che precede il botto finale della finanziaria più spietata degli ultimi dieci anni, compresi quelli dei cinque Governi di centro-sinistra. Tali Governi, sia pure nel balletto verde-rosa della legislatura precedente alla precedente, mai hanno osato parlare il linguaggio cinico e baro

Delle clientele della sinistra? Dei carrozzoni che non smantellate o che perfezionate, ammantandoli della definizione elegante dello *spoils* *system*, che significa cacciare quelli che c'erano prima e mettere tutti i vostri, come ha fatto la simpaticissima ministra Turco, presente in Aula a sfidarci coraggiosamente? La Ministra ha sostenuto che ha cambiato un oncologo con un altro; mentre tutto il centro-destra la attaccava, io l'ho difesa, perché ritengo che un Ministro abbia il diritto di esercitare le sue competenze. Ma la signora Turco, molto poco gentilmente, ha sostituito tutto il Consiglio superiore della sanità

Ma il sospetto delle vostre scelte, che questa manovra finanziaria autorizza e conferma, è che chiediate i soldi per aggiustare le clientele e il fiato grosso della piazza, dei sondaggi, del Paese che si ribella non vi trasmette il germe del dubbio, ma, al contrario, aumenta i vostri appetiti, perché vi sentite convitati di una tavolata che volge al

che prende insieme la finanziaria ed il collegato fiscale, si è discusso molto su singole misure, su presunti o effettivi aggravi fiscali, ma poco, pochissimo delle vere ragioni degli obiettivi della manovra finanziaria, di cui il provvedimento in esame è parte integrante. Nutriamo, infatti, la speranza che il Paese, l'economia possano ripartire dopo anni di stallo. Nell'anno corrente ci aspettiamo una crescita, dopo anni di essere stati fermi sullo zero per cento della crescita del PIL. Speriamo di arrivare all'1,7 o al 2 per cento a fine anno, ma non dimentichiamoci che il resto d'Europa è già partito e ci supera di gran lunga; la Grecia: più 4, 3; la Spagna: più 3, 8; la Germania: più 2, 8 e potrei proseguire, ma la faccio breve: la media dell'Unione Europea è al 2, Pesano, infatti, sulla nostra economia due grandi problemi strutturali che frenano la crescita: il primo è l'indebitamento dello Stato, il secondo la relativa bassa produttività delle imprese. Il Governo intende fronteggiare entrambi i problemi con risolutezza, con una graduale riduzione del debito pubblico e tramite misure di liberalizzazione. Vorrei fare un brevissimo *flash* sul passato: abbiamo avuto negli anni novanta un disavanzo pubblico annuale che andava oltre il 10 per cento annuo; abbiamo poi stupito l'Europa a metà degli anni con il risanamento dei conti pubblici che abbiamo portato sotto la misura di Maastricht del 3 per cento, addirittura nel 2000 allo 0,6 Purtroppo, dal 2001 in poi, il debito ha cominciato a crescere e così l'indebitamento netto dello Stato annualmente per sforare per la prima volta già nel 2001, con il nuovo Governo Berlusconi, il 3 per cento, arrivando adesso probabilmente al 4, 6 per cento di quest'anno. Ed il debito pubblico complessivo - di cui si sta parlando - ha raggiunto la cifra astronomica di 1.400 miliardi di euro. Stiamo parlando di un bilancio di 40 miliardi di fronte ad un debito pubblico di 1.400, che costano ai contribuenti 65 miliardi di interessi annui: 65 miliardi è ben oltre di quanto è questa misura finanziaria! Difatti, siamo stati declassificati dalle aziende

Pertanto, per tutte le critiche piovute su questo Governo, devo chiedervi: l'economia, le imprese devono essere le prime interessate a far crescere e ricrescere nuovamente questo Paese fermo o vogliamo indebitarci ancora di più e fare come una famiglia che spende tutti soldi per pagare gli interessi alla banca? Pertanto, l'obiettivo centrale di questa manovra è la ripresa del Paese ed il rilancio dell'economia. L'obiettivo è quello di liberare risorse per favorire la crescita e lo sviluppo. Difatti, è stata approvata con lode la manovra dalla Commissione di Bruxelles, dalla Banca centrale di Francoforte e dal Fondo monetario internazionale che hanno approvato l'obiettivo di scendere con il *deficit* pubblico sotto il 3 per cento, allineandoci a quanto prescrive l'Unione Europea.

ed è la seguente. All'inizio del dibattito sulla finanziaria il Governo avrebbe dovuto dire al Paese a chiare e tonde lettere in quale situazione catastrofica ci troviamo

assumere misure che costano anche dei sacrifici ai cittadini. Questo aspetto è stato forse nascosto troppo, ma è giusto che sia evidenziato perché questa era la scelta dovuta da fare che forse avrebbe portato meglio, in particolare i settori economici che hanno lamentato gli aggravi. Dovevamo inoltre dire che, grazie all'impegno

risolte le questioni dello scontrino fiscale e dell'ammortamento degli immobili strumentali (sono modifiche importanti) e dell'esonero del settore agricolo per quanto riguarda

nel presentare gli emendamenti alla finanziaria qui in Senato. Ricordo il patto tra fisco e contribuente e il rispetto dello Statuto del contribuente, l'impegno di rivedere il regime fiscale degli autoveicoli e l'impegno di destinare le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale alla riduzione della pressione fiscale

Rimane soprattutto, onorevole Presidente, l'obbligo di far seguire riforme strutturali, che coinvolgano tutto il settore dell'apparato burocratico, della pubblica amministrazione (dove i risparmi sono ancora possibili), dell'energia e della previdenza.

Auspichiamo - dicevo - lo sviluppo del federalismo fiscale, al fine di trasferire alle Regioni e alle Province la responsabilità non solo per le uscite, ma anche per le entrate. Le stesse verrebbero così responsabilizzate maggiormente e ciò favorirebbe la lotta all'evasione fiscale. Riassumendo: condividiamo l'obiettivo di ridurre il debito pubblico per rilanciare il Paese, fermo da ormai troppi anni; accogliamo con favore le modifiche finora apportate e, fiduciosi che il Governo vorrà recepire nella legge finanziaria per l'anno 2007 le proposte migliorative che presenteremo come Gruppo Per le Autonomie, annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo su questo provvedimento. *(Applausi

Italiani. In premessa, credo che la maggioranza abbia raggiunto un risultato politico importante. l'iniziativa dell'opposizione, che ha tentato in qualsiasi modo, in queste ore, di costringere il Governo a porre la fiducia, per dimostrare che questo ramo del Parlamento sarebbe ingovernabile senza le successive richieste di voti di fiducia. L'opposizione è stata L'opposizione è stata sconfitta dalla compattezza della maggioranza. Credo si tratti di un successo politico importante, ma soprattutto della dimostrazione della condivisione profonda, da parte della maggioranza, dei contenuti del provvedimento che

Presidente, colgo l'occasione di questo intervento anche per esprimere profonda solidarietà nei confronti dei senatori a vita, che sono stati attaccati in queste ore in modo pretestuoso e smodato. hanno solo esercitato il loro diritto costituzionale a votare, come prevede la nostra Costituzione. Si preannuncia in queste ore, da parte della destra, un'iniziativa di riforma costituzionale per impedire ai senatori a vita di esercitare questo diritto. Noi non saremo mai d'accordo su questa iniziativa; ma, soprattutto, non siamo d'accordo adesso, perché risulta un'iniziativa astiosa, vendicativa, intimidatoria nei confronti dei senatori a vita,

a vita non tanto per il loro voto, che hanno esercitato secondo quanto prevede la Costituzione, quanto per la loro presenza insieme a tutti noi, maggioranza e opposizione, in queste ore di lavoro intenso. Gli assi fondamentali del provvedimento sono la lotta all'evasione e all'elusione fiscale e il recupero di base imponibile; misure in netta discontinuità con il passato Governo. C'è differenza tra la lotta all'evasione e i condoni tombali; sono scelte radicalmente alternative. Il condono tombale sana i contenziosi fiscali, sana i contenziosi amministrativi e penali e garantisce l'impunità e l'anonimato. Quello che si è verificato lo abbiamo visto in queste settimane: chi ha condonato ha pagato la prima rata e poi è rientrato nel nero.

efficaci, sono vigenti in altri Paesi europei che sono democratici; altro che Stato di polizia. Noi vogliamo veramente fare la lotta all'evasione fiscale, è per questo che votiamo a è anche per questi motivi che il nostro Gruppo sostiene con forza e convinzione questo provvedimento. *(Applausi

onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghe e colleghi, innanzitutto vedo che il Sottosegretario si complimenta. Ha ragione anche il senatore Ripamonti: la maggioranza ha tenuto; non solo, la spallata non c'è stata, il fortino il fortino della maggioranza ha retto, anche con i nuovi soldati, cioè i senatori a vita cui vanno i complimenti per la tenuta fisica. Vorrei che le nuove generazioni avessero questa tenacia, ma purtroppo, cominciando dalla mia, non abbiamo

La maggioranza aveva affermato che in questo Paese bisognava riformare la ricerca, investire nella ricerca. Certo, l'investimento c'è stato, onorevoli colleghi, prima di tutto da parte dei vari Pistella che, lo ricordo, sono persone arrivate da voi in qualche modo e sono al di sopra delle parti.

quelli che ormai avete criminalizzato; qui, infatti, c'è un odio comunista di classe. Presidente Marini, vi siete alleati e alla fine avete trovato la quadra in un odio comunista di classe contro il commerciante,

come fa il presidente Benvenuto: come si fa a dire che si è triplicato il lavoro nero con il Governo Berlusconi? Dà i numeri. Abbiamo avuto 28 miliardi nuove entrate, un nuovo rapporto con i contribuenti fiscali; fiscali; c'è stata un'emersione del lavoro nero. I cosiddetti lavoratori Co.Co.Co., ricordiamolo, i lavoratori precari vi servono per andare in piazza e bruciare i fantocci.

e che voi sottoponete ai criteri di Visco. Provate a chiedere agli artigiani che votano per voi, o alla classe media, cosa pensano di Visco. Se potessero dargli un voto, non arriverebbe a Questi non sono delinquenti, ma persone che hanno fatto l'Italia, la Padania. Allora voi gli mandate i Carabinieri, gli mandate gli accertamenti fiscali e gli agenti occhiuti di Visco;

Quindi, restate pure nel fortino. Stasera festeggiate questa vittoria sulle mura. Festeggiate anche con i giovani rampanti che si sono prestati a un voto disciplinato. È stato disciplinato, complimenti. Poi provate a andare in giro

fin dal primo giorno della legislatura abbiamo presentato un progetto di riforma per rivedere le norme sulla contabilità perché il «mostro» che sta per arrivare sulla finanziaria è diventato qualcosa di incontrollabile e ingestibile. Il Paese non può reggere uno *stress* così dannoso. Questo decreto-legge, con scelte maturate fuori da ogni logica di concertazione, è il frutto avvelenato di veteromassimalismo e pansindacalismo, neppure coniugato con finto liberismo. Nelle vostre risposte c'è qualcosa di arcaico. Riportate il Paese indietro nel tempo, ad un sessantottismo al potere che rivendica un doppio ruolo: quello di lotta e di governo. Protestate e marciate contro le vostre stesse scelte. Altro che sostituzione di pezzi di maggioranza! Questa è una manovra falsa e sbagliata. Falsa sull'entità delle cifre contrabbandate, sbagliata nella qualità e nella quantità degli interventi. Manovra eccessiva, iniqua, ostile alla crescita e con pochi tagli sulla spesa: è il giudizio di Fiorella Kostoris, *ex* Padoa-Schioppa, che non abbiamo mai visto in quest'Aula. E' stata bocciata non solo dalle agenzie di *rating*, ma dai corpi sociali, dai settori produttivi e dalle categorie economiche. Avete infierito pesantemente contro i ceti medi produttivi nelle nuove articolazioni dopo il processo di terziarizzazione, fisiologica dinamica di un capitalismo maturo, e soprattutto contro il sistema della piccole e medie imprese e quelle artigiane, quei comparti che sono la ricchezza produttiva del Paese. I dati sul gettito fiscale e l'andamento del fabbisogno di cassa hanno smentito clamorosamente i risultati della commissione Faini e il vostro catastrofismo, proteso a creare un'illusione finanziaria per soddisfare le richieste della coalizione che ha imposto una dilatazione della spesa pubblica per 13 miliardi di euro, contrabbandata per misure allo sviluppo. Avete espropriato il TFR. Vi accingete alla riforma del catasto. Non si affrontano i nodi strutturali del Paese, né le vaste aree di spreco, preferendo introdurre nuovi balzelli, puntando sull'aumento della entrate fiscali, dirette, indirette e contributive, con una grandinata di balzelli che faranno innalzare la pressione fiscale di due punti. L'evasione fiscale per noi non è un mero proclama, ma una cosa seria che richiede strumenti seri. Noi non difendiamo gli evasori. Non c'è alcuna giustificazione morale nei loro comportamenti. Un fenomeno così diffuso si affronta in modo serio ed efficace con lo strumento principe che è quello del contrasto di interessi, recuperando un clima di fiducia tra cittadino e Stato. Va resa detraibile una serie di operazioni per la famiglia e per la casa. Non è, dunque, ministro Padoa‑Schioppa, un adempimento fastidioso per i contribuenti. Che dire, poi, degli scontrini fiscali, su cui abbiamo assistito ad un balletto interparlamentare di posizioni contrastanti? Avete una visione obliqua della società; avete posto la definizione di ricco dentro un parametro ingiusto e incomprensibile: un'analisi che dia impostazione esclusiva o prevalente alla quantità è monca e fuorviante, avrebbe detto Paolo Sylos Labini; avete voluto colpire il ceto medio, che non è un artificioso recinto statistico, ma è, invece, costituito da coloro che cercano una propria base di lavoro per sviluppare una propria attività con vecchie e nuove professioni. Onorevole signor Presidente, con le vostre scelte avete messo a rischio le prospettive di crescita dell'economia: non è una manovra che fa alzare tutte le barche, ma solo quelle della rottamazione, dei settori maturi e dei molti amici di questa maggioranza. Vi è, invece, il pericolo che molte affondino, preferendo il mare aperto della delocalizzazione piuttosto che affondare nello *tsunami* del vice ministro Visco. Lasci agli storici, il ministro Di Pietro, il compito di valutare la storia, signor Presidente, che è una storia di crescita sociale, economica e di grande progresso nella libertà. Pensi, piuttosto, alla figura cui ha esposto il Paese con la doppia palese infrazione comunitaria e le sue scelte in materia di concessioni autostradali. State mettendo a rischio il programma di opere pubbliche, soprattutto per quelle grandi direttrici europee (la Torino-Lione e la Palermo-Berlino) essenziali per lo sviluppo del Paese. Signor Presidente, mi avvio alla conclusione: non vi è una funzione politica di educazione del contribuente; non vi è quell'impronta vanoniana

Il Presidente del Consiglio Prodi si è assunto una grave responsabilità nell'avere costruito un cartello elettorale disomogeneo incapace di governare, di assumere decisioni coerenti nell'interesse del Paese inseguendo un consenso che non c'è e non potrà esserci. Purtroppo le vostre decisioni sono funzionali alla maggioranza ma non per il Paese perché le vostre "illusioni finanziarie" dilatano la spesa e rischiano di soffocarne le prospettive di crescita con una manovra di bilancio contraddittoria, classista, odiosa, dannosa e inutile.

sarò molto breve e, eventualmente, consegnerò alla Presidenza l'argomentazione del

- contrariamente a quanto si può intendere dalla sua rappresentazione in Aula - non possiamo dimenticare il fatto che un confronto di merito sulle questioni, anche registrando interlocuzioni

che la maggioranza non avrebbe promosso emendamenti al provvedimento in esame, alla luce di un ragionamento molto semplice e molto lineare. Questo provvedimento si configura come lo strumento per dare copertura finanziaria per circa 7 miliardi di euro alla finanziaria. Quindi, esso s'inserisce in un meccanismo complessivo della manovra che il Governo

Sulla base di questo, per altro, si è provveduto ad un confronto serrato anche con il Governo, oltre che tra le forze politiche, traducendo in una serie di ordini del giorno, accolti dal Governo, indicazioni che derivano anche da valutazioni critiche rilevate su questo provvedimento. È noto che la nostra impostazione di una manovra economica l'avremmo preferita diversa; non ne abbiamo fatto mistero. tuttavia, puntato comunque ad una manovra che avesse un equilibrio forte tra risanamento, equità e sviluppo. Questo penso che ci sia; certo, se si pensa che questo possa rappresentare una sorta di costruzione di una società da «Grande fratello» di orwelliana memoria per il semplice fatto che si chiede e si propone di organizzare un sistema che in tutti i Paesi democratici, di democrazia liberale e di economia capitalista, è diffuso ed è sistema corrente,

Tecce e Albonetti che sono intervenuti nel merito - che abbiamo accettato coerentemente la sfida di contribuire a realizzare gli obiettivi che nel programma dell'Unione ci eravamo prefissati. Questi obiettivi continueremo a perseguirli anche nella fase di discussione della finanziaria e sono convinto che che il segnale che il Governo ha inteso recepire in sede di Commissione, ancora di più debba impegnarlo responsabilmente a interloquire positivamente anche nella fase di discussione della finanziaria.

nell'annunciare il voto contrario del Gruppo di Alleanza Nazionale, vorrei brevemente svolgere una premessa e quattro motivazioni. La premessa è che l'opposizione, molto responsabilmente, ha tentato di far entrare in quest'Aula un confronto e un dibattito nel merito del provvedimento. Nonostante questo, tale dibattito non c'è stato, perché, come si usava un tempo nelle vecchie classi elementari, quando la classe si agitava troppo e faceva confusione, il maestro interveniva e lanciava ai bambini l'idea di fare il gioco del silenzio. Immediatamente la classe taceva, anche perché il primo che parlava perdeva il diritto ad avere la merendina durante la ricreazione. Ebbene, cari colleghi della maggioranza, avete fatto il gioco del silenzio. Il fatto di non aver posto la questione di fiducia è stato sopravanzato dal vostro silenzio dirompente nel merito nei contenuti della manovra. Non era questo, evidentemente, l'obiettivo dell'opposizione, ma quello di avere un pacato, sereno, serrato confronto nei contenuti; prendiamo atto che ciò non è avvenuto.

ha intrapreso un gioco di singoli individui e ha scelto il pugilato contro l'economia e la società italiana. Un pugilato fatto di tre colpi e, ovviamente, ogni volta, si manda sul *ring* il personaggio della maggioranza che ha il muso più duro. Il primo, diretto al mento, è stato sferrato all'economia e alla società italiana con il cosiddetto decreto Visco-Bersani. Il secondo, gancio sinistro, è quello che vi apprestate a votare con questo decreto-legge. L'*uppercut* finale che stenderà ko l'economia e la società civile italiana è la legge finanziaria, che vi apprestate a votare, con molta probabilità anche in questo caso, con il voto di fiducia o con il gioco del silenzio imposto dal maestro furbacchione. Sarebbe ora di smetterla di attribuire al precedente Governo lo sfascio dei conti pubblici e un'economia sull'orlo del precipizio. Sarebbe opportuno che parlaste un po' di più con il vostro Ministro dell'economia, che scrive ufficialmente nei suoi documenti che complessivamente la vostra legge finanziaria, includendo questo decreto fiscale, solo per 15 miliardi di euro al risanamento dei conti pubblici. E voi della maggioranza vi dovreste chiedere perché una manovra di risanamento di tale entità diventa una manovra di oltre 40 miliardi di (quasi 45 miliardi, se sommiamo i 6 miliardi del decreto Visco-Bersani di luglio che hanno effetto esclusivamente sul 2007). La risposta è molto semplice: semplice: si gravano gli italiani di 30 miliardi di tasse per portarle dentro i portafogli di alcuni Ministeri, per accentrare il potere economico e civile

non è una legge finanziaria quella che state votando, ma una manovra di accentramento di potere economico e civile, condita da due reati:

basta fare i conti con i numeri del Governo. Con questa finanziaria il *deficit* pubblico, correttamente calcolato secondo le regole della contabilità dello Stato, l'anno prossimo rischia di sfiorare il 4 per cento rispetto al prodotto interno lordo.

dall'Eurostat conti che sono contrari alla contabilità dello Stato. Basta ricordare che nel 2001 l'Eurostat certificò un *deficit* dello 0,8 per cento e due anni e mezzo dopo lo stesso Eurostat dichiarò, come dai dati ufficiali, che il *deficit* era del

che taglia lo sviluppo, introduce più iniquità fiscale e non raggiunge le condizioni di equilibrio finanziario. *(Applausi

nel preannunciare il convinto voto contrario di Forza Italia voglio fare alcune premesse. Non entrerò negli aspetti tecnici, che sono stati più volte ripetuti,

Voglio ricordare che la teoria del ciclo economico-politico, elaborata da Nordhaus molti anni fa, si fonda sull'ipotesi che i politici massimizzino la probabilità di essere eletti, oppure rieletti, e che i partiti si comportino in modo opportunista, cioè manipolando le scelte egli elettori, sfruttando i loro difetti di informazione. Il ciclo politico economico di Nordhaus non nasce come effetto secondario di politiche aventi altre finalità, ma è il risultato dell'ipotesi che le decisioni dei politici siano espressione delle loro preferenze proprie.

prossima, determinino un maggior aggravio fiscale che non sarà solo ed esclusivamente determinato dalla finanziaria, ma da tutti gli effetti di amplificazione di Comuni, Province e Regioni che sfiorano sfiorano i 50 miliardi di euro. Stiamo ponendo chiaramente le premesse per tale impostazione. Del resto, il presidente Prodi ha detto: i primi sei mesi facciamo così e poi avremo tempo di redistribuire.

che occupava 260 pagine di *Gazzetta Ufficiale*, partita con 76 articoli e arrivata a 158, che prevedeva

ipoteca per l'operato del Governo Berlusconi. E voi avete oggi la faccia tosta di ricordare alcuni aspetti di catastrofismo che erano solo ed esclusivamente delle bugie elettorali, perché ricordo che la commissione Faini ha certificato che il Governo Berlusconi ha ben operato. Ho ascoltato i relatori riproporre le lamentazioni sulla crescita della percentuale di spesa corrente sul PIL avvenuta negli ultimi anni, come se potessero ignorare, seguendo l'analisi economico-politica con la quale ho esordito, ovvero questa teoria che voi state mettendo in perfetta funzione, funzione, un elemento da prime pagine di economia: il fatto che non si può o risulta estremamente difficile comprimere la spesa corrente nelle fasi di bassa crescita, pena l'ulteriore aggravamento e ripiegamento ciclico dell'economia rispetto alle fasi positive di crescita del prodotto. *(Richiami del Presidente)*. In queste vostre angolazioni, non tendete alla necessità di un forte recupero della produttività e il risanamento - lo ricordo - si ottiene agendo più sulle spese e meno sulle entrate e sui risparmi. State portando avanti un blocco culturale dove non fate altro che incrementare, in una base ideologica, il consociativismo, il cooperativismo e il metodo di cooptazione.

che tutti i maestri dell'economia (cito Vilfredo Pareto per tutti) scrivevano, e scrivono - e i fatti storici ci danno ragione

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho scelto di parlare senza iattanza, ma è solarmente evidente che oggi l'Unione e il Governo registrano qui al Senato un grande risultato politico e - lasciatemelo dire - il più significativo dall'inizio della legislatura. *(Applausi Esso non è il frutto di una contingenza numerica di presenze, è il frutto di una decisione politica che abbiamo convintamente perseguito voto per voto (87 nelle ultime due giornate), a partire da martedì della scorsa settimana, dai giorni in cui, prima sui presupposti di costituzionalità, poi sulle pregiudiziali, poi ancora, da ultimo, sulla richiesta di non passaggio all'esame degli articoli, l'opposizione annunciava la cosiddetta spallata al Governo. Una decisione politica che è riuscita a non lasciarsi inquinare dalla tentazione della contrapposizione muro contro muro, dalla tentazione di ricorrere al voto di fiducia, strada che sarebbe stata pienamente legittima - lo voglio ribadire - e che tante volte il Governo Berlusconi, in circostanze analoghe, con ben altre maggioranze, invece ha scelto. Abbiamo scelto la strada più aspra, difficile e rischiosa di consentire che qui al Senato - come è giusto che sia - le ragioni dell'opposizione avessero piena espressione e che si potesse celebrare qui il più sacro dei riti della democrazia: la comunicazione compiuta al Paese delle ragioni di chi dissente, anche dei colleghi che di coloro che nutrono dissenso e critica nei confronti della maggioranza, nei confronti di chi governa. In qualche modo, colleghi dell'opposizione, noi tutti, Capigruppo della maggioranza e senatori, che ringrazio tutti davvero di cuore, abbiamo contribuito con sacrificio e con rischio e lo abbiamo fatto su un testo blindato per la necessità di consentire al Paese di vedere completata la manovra di bilancio Vedete, colleghi, l'abbiamo fatto - non vorrei usare parole grosse - anche per voi; e per questa ragione, innanzitutto, giudico un errore politico l'aver qui sollevato, sia pure nei modi con cui l'ha fatto ieri il presidente Schifani (gliene do atto), la questione del diritto di voto dei senatori a vita, perché inevitabilmente, in questo contesto, essa appare come frutto di rivalsa politica, figlia di acrimonia, cifrata da vendetta.

il mio Gruppo non cesserà di lavorare perché l'essenza della democrazia moderna, la ricerca di soluzioni condivise sulle questioni strategiche per il Paese e per il suo futuro trovino qui, al Senato, la possibilità di inverarsi. Altro che Governo di larghe intese! Noi stiamo ragionando del superamento della transizione italiana, della fondazione di un bipolarismo maturo, più attento agli interessi generali del Paese che alle alchimie che appassionano certi commentatori politici. Un'ultima considerazione, colleghi. Ieri la rappresentazione che è venuta a me e a tanti colleghi (direte parziale; è possibile, il Paese ci dirà come l'ha vissuta) del lungo dibattito sull'ordine del giorno presentato dal senatore Schifani, dibattito attuato peraltro con generosa disinvoltura rispetto al Regolamento, è apparsa più come una disputa delle forze di maggioranza intorno al simbolismo del ponte. Altrimenti non capiremmo, vice presidente Baccini, gli attacchi francamente ingenerosi e altrimenti inspiegabili che le sono stati mossi, come se ciascuna forza politica della Casa delle Libertà dovesse qui disputarsi un simulacro. Questo decreto destina alla Sicilia...

o non vuole intenderlo - celebra il ruolo del Senato, assicura il Paese circa l'esistenza di una classe dirigente che continuerà a lavorare assumendosene la responsabilità, per tirarlo fuori dalla lunga transizione italiana.

dovevo votare contro e invece ho votato a favore. Signor Presidente, sono parlamentare di abbastanza lunga data per sapere come i vecchi strumenti di controllo parlamentare (interrogazioni e interpellanze) abbiano perduto ormai ogni valore. Sarei qui a sollecitare la risposta a circa quaranta, tra interpellanze e interrogazioni, ma sono abbastanza vecchio per sapere che il Governo alle interrogazioni e alle interpellanze non risponde mai.

Per suo conto ha risposto lo scagnozzo di quel losco figuro del capo della polizia che si chiama Gianni De Gennaro. Questa è un'offesa a me? Gianni De Gennaro ha una tale bassezza morale che non mi può offendere neanche se mi sputa in faccia. Un uomo che è passato indenne da manutengolo della FBI americana, è passato indenne dalla tragedia di Genova, è passato indenne dopo aver confezionato la polpetta avvelenata che ha portato alle dimissioni di un Ministro dell'interno; è passato indenne da tante cose. Però, mi dispiace per il ministro Amato,

buona memoria di ciò che ha richiesto. Va da sé che i giudizi che sono stati espressi sul capo della Polizia ovviamente appartengono

***Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di ritenere che le dichiarazioni per

lei giustamente non può conoscere questa informazione. Occorre poi considerare che a quella seduta non ha partecipato nessun membro dell'attuale maggioranza, proprio perché si stava svolgendo in quella delicata giornata un confronto interno alla stessa, che è stato conseguenza

e non c'è stato verso di far sospendere la riunione della Giunta. Ora, signor Presidente, non so come ella intenda proseguire i lavori su questo punto,

Quindi, è importante che i colleghi senatori comprendano bene la valenza dell'uno e dall'altro procedimento di richiesta di autorizzazione a procedere.

solo dire che la ricostruzione del collega Lusi è parziale e inesatta. In quell'occasione vi era effettivamente questa riunione della maggioranza, ma io ricordo perfettamente, essendo membro della Giunta e avendo partecipato ai lavori anche in quella seduta, che i componenti della Giunta appartenenti ai Gruppi di maggioranza

che si sia assunta una decisione in loro assenza non è stato certamente dovuto a una prevaricazione o a un voler approfittare di una situazione, visto che loro erano tutti lì e potevano entrare e votare, così come abbiamo fatto noi. [DI

l'unanimità di quella seduta era una unanimità dei presenti e non l'unanimità della Giunta nel suo complesso. Le questioni sono due e attengono entrambe alla facoltà che il senatore Iannuzzi si riconosce di scrivere e di acquisire, anche nella sua veste di giornalista periodista, la qualità di senatore. Quindi, il problema non è tanto (intervengo nel merito)

in un processo su questo sindacalista Geraci della CISL ucciso e, per un'altra procedura, su dei su dei pubblici ministeri di Palermo. Non è questo l'oggetto del nostro voto: l'oggetto del nostro voto è se il senatore Iannuzzi in questa sua veste di giornalista abbia esplicato anche le funzioni di senatore, e noi crediamo che le funzioni di senatore non possano essere richiamate per un'attività che tra l'altro Lino Iannuzzi svolge anche con contratti giornalistici. Ripeto: se si trattasse di un giudizio di un giudizio di merito processuale forse sarei il primo a dire che non c'è materia del contendere, che non bisognerebbe nemmeno procedere, perché sono giudizi che attengono ad una sua valutazione, alla libertà di espressione. Però, il problema qui è che noi abbiamo un potere molto limitato: noi dobbiamo solo stabilire se quelle affermazioni siano state fatte come

se debba essere rinviato o meno a giudizio per questa ragione. Il nostro giudizio è che purtroppo noi siamo quasi obbligati, almeno come Rifondazione Comunista, a votare contro la decisione della Giunta, anche perché esiste una lunga giurisprudenza della Corte costituzionale,

ha sempre accolto il conflitto di attribuzioni sollevato dalla magistratura e ci ha sempre dato torto. Quindi, se si vuole

l'altra strada, che non è stata sollevata formalmente e a cui mi pareva alludesse l'intervento del senatore Lusi, è una richiesta di sospensione,

Presidente, credo che la richiesta del senatore Lusi, anche se non ancora formalizzata, debba essere valutata attentamente. Si tratta di due questioni particolarmente delicate, che riguardano un senatore della Repubblica a causa di affermazioni rese in un contesto particolare e in funzione delle quali la Giunta si è espressa in un certo modo. Do atto al senatore Lusi che la decisione è stata adottata all'unanimità dei presenti, anche perché è difficile coinvolgere nell'unanimità gli assenti. L'unanimità è sempre dei presenti, chi c'era si è espresso unanimemente a favore dell'insindacabilità. È chiaro che chi non c'era non poteva esprimersi. Ritengo, quindi, che per questi due casi così particolarmente delicati, dopo dei lavori di Aula che hanno tenuto impegnati i senatori nella giornata di ieri e nell'intera mattinata di oggi,

di questa Assemblea. Per quanto mi riguarda, aderisco alla richiesta del senatore Lusi.

la proposta di modifica del Regolamento del Senato volta ad istituire la 15a Commissione permanente sui diritti delle donne e sulle pari opportunità, che ricalca strutture

una gentile concessione da parte del Governo e della maggioranza, perché l'ordinario svolgimento dei lavori prevede che non si apponga la fiducia e dunque che le Camere, in particolare il Senato, facciano il loro dovere di legislatori, come previsto dall'articolo 70 della Costituzione. Costituzione. Non so se il non aver apposto la questione di fiducia dipenda dal fatto che non si capisce quali siano le modalità con cui questo Governo decide di apporre la questione di fiducia. Per la quinta volta, dunque, sollecito la risposta alla mia interrogazione, che riguarda i modi e i tempi misteriosi con cui fu decisa, da parte del Consiglio dei ministri (perché non risulta possa essere presa da altri organi), l'apposizione della questione di fiducia sul cosiddetto decreto Bersani l'ormai lontano 25 luglio. Si riunì il 21 luglio - data, peraltro, foriera di terremoti istituzionali - il Consiglio dei ministri, ma non decise nulla, per esplicita affermazione del segretario del Consiglio dei ministri, onorevole Enrico Letta,

che il giorno domenica 19 novembre ho inviato una lettera al presidente del Senato, Franco Marini, nella quale chiedevo che una sala del Senato della Repubblica fosse intitolata ai caduti di Nasiriya.

ricordarli intitolando una sala di questo Palazzo delle istituzioni a quei nostri militari, forse da qualcuno dimenticati*.

che la giornata del 25 novembre è dedicata dalle istituzioni internazionali alla violenza contro le donne. Mi associo quindi alle sue parole, a nome non solo delle senatrici, ma di tutto il Gruppo di Rifondazione Comunista.

pensano di poter risolvere con la violenza i conflitti che all'interno della famiglia, del mondo del lavoro e delle relazioni tra i sessi possono nascere. È agli uomini che È agli uomini che dobbiamo porre interrogativi, perché sono loro che devono darsi, con l'aiuto delle istituzioni, risposte sul perché rispondano in questa maniera ai conflitti di genere. Mi associo anche a quanto sostenuto dalla senatrice Negri

iniziative volute da istituzioni locali, da associazioni di donne e, soprattutto, dai centri antiviolenza, per ricordare e combattere questa piaga che attanaglia la nostra come molte altre società.

insisto e ribadisco la riflessione di ieri al Senato, per portare alla Giunta per il Regolamento o per formalizzare comunque un *iter* di modifica regolamentare in relazione al ruolo dei senatori a vita.

La novità politica è che per la prima volta il centro-destra andava oltre i 156 voti e quindi allargava la sua potenzialità e la sua forza e, dall'altra, la conferma che, ancora una volta, i cinque senatori a vita sono stati determinanti.

ossia alla necessità di favorire rapidamente l'*iter* di quelle proposte che vanno nel senso di insediare presso la nostra Camera e presso il Senato una Commissione che, al pari di tutti gli altri Paesi, lavori con costanza e coerenza per l'affermazione dei diritti delle donne e per le pari opportunità - ricordo che il 2007 è per l'Europa l'anno delle pari opportunità così come anche l'importanza di essere coerentemente impegnati su temi sui quali tutte le nostre Regioni e altre istituzioni europee internazionali lavorano e rispetto ai quali indubbiamente, dal punto di vista dei nostri strumenti strumenti di lavoro, siamo in questo momento carenti. Ritengo anche che sarebbe opportuno un impegno di questa Assemblea, entro la fine di quest'anno, a ricordare e a e a celebrare l'evento della conquista del voto per le donne; un evento tardivo nel nostro Paese, a tal punto tardivo che ancora oggi siamo qui a combattere per affermare il diritto ad una cittadinanza piena e la parità